PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Assistiamo a celebrazioni un po' auliche, e probabilmente fuori tempo, della visita di un dittatore che calpesta i diritti umani nel suo Paese

*IdV)*. Non si può trattare quest'Aula come se fosse una sala stampa o un cineteatro. Qui non si recita nessuna commedia! commedia! Insisto, noi passeremo a forme di protesta eclatanti a difesa del Parlamento

se il Governo italiano sta insistendo così tenacemente, vogliamo sapere cosa c'è sotto, realmente, per Parlamento. Può andare in qualsiasi altra sala pubblica per parlare, ma non nel nostro Parlamento, che è un baluardo di democrazia.

è il ruolo del Parlamento; a volte, infatti, partendo dall'intenzione di difendere il ruolo e il prestigio del Parlamento, si può determinare

Signor Presidente, colleghi, sarò veloce nell'analisi della legge comunitaria. Voglio tuttavia

Questa legge si scontra con due problemi fondamentali, e il fatto che si sia già in terza lettura lo dimostra. Il primo problema è rappresentato

Perfino il Ministero dell'interno greco, che per anni ha dato i nomi degli amministratori locali, non lo fa più. C'è poi l'articolo 10, in cui si parla dell'inquinamento nella Pianura padana. Poiché la Pianura padana è italiana, e non appartiene ad un solo Gruppo parlamentare,

CCISS-Viaggiare informati e di Isoradio, che fanno veramente un servizio pubblico. Sull'articolo 45, come ho detto, interverrà il collega Vita. Voglio ora esporre al ministro Ronchi, ai colleghi della maggioranza e ai colleghi che hanno partecipato alle elezioni europee una brevissima riflessione. Questa legge deve inquadrarsi in una riforma che riguarda l'Europa e le sue istituzioni. Noi abbiamo bisogno di un'Europa che sia fatta di politiche dell'Unione europea e non di pause di riflessione, che hanno portato a due *referendum* persi in Francia e in Olanda e poi a quello in Irlanda.

e mi rivolgo anche a noi, che abbiamo riportato la prima presenza per numero di voti nel raggruppamento dei riformisti europei e la seconda per numero di parlamentari europei. Credo che dobbiamo impegnarci per un mandato costituente,

ma anche e soprattutto perché sia superata la Conferenza intergovernativa e sia convocata una nuova Convenzione per dare una Costituzione all'Europa e per fare in modo, come hanno affermato il presidente Napolitano e il presidente emerito Ciampi, che l'Europa sia fatta con coloro che vorranno farla. Bene, speriamo che in questa Europa - oltre che con la legge comunitaria, che è un obbligo - l'Italia ci sia. Purtroppo, malgrado l'impegno anche del ministro Ronchi, questo dato non è sicuro. Noi faremo la nostra parte: sappiamo che il Partito popolare europeo, la casa che alcuni di noi hanno costruito, ma che abbiamo lasciato perché ormai divenuta la casa dei conservatori, ha comunque basi europeiste. Siete voi della maggioranza che dovete corrispondere alle attese che riguardano l'Europa. Noi vi diamo appuntamento in Europa, rivendichiamo l'Europa dei padri fondatori, ma anche quella di Delors, di Mitterrand, di Kohl, di Romano Prodi e di Ciampi. È un appuntamento alla politica quello che vi diamo. Noi - le donne e gli uomini del PD, i militanti e i parlamentari europei, gli 8 milioni di voti che il Partito Democratico ha riportato - in Europa ci saremo. Vi aspettiamo: è un appuntamento alla politica che speriamo non vorrete mancare.

pongo, anche a nome di altri colleghi, un tema recente, ma molto più antico nelle sue premesse, segue: il passaggio dalla tecnica di diffusione radiotelevisiva analogica, che ci ha accompagnato per almeno un cinquantennio, a quella digitale potrebbe essere una straordinaria occasione per un Paese come il nostro, che ha ancora tante arretratezze,

è l'occasione per riaprire le coordinate generali del sistema; è la premessa per ricostruire un'industria culturale, che in Italia è entrata via via in difficoltà, anche dopo i tagli apportati alla spesa culturale,

all'inizio degli anni Novanta, di accelerare in Italia - non per caso - il passaggio al digitale, fu anche per stimolare un'opportunità industriale che sembrava sepolta. Siamo al dunque. L'articolo 45, purtroppo, ci sembra una ben misera risposta a queste grandi opportunità, in quanto si dà sostanzialmente legittimazione ad un atto che è stato discusso anche con diverse contrarietà, espresse in modo molto argomentato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; un atto che certamente il tema di cui stiamo discutendo. In sostanza, l'articolo 45, come ha detto bene il collega Di Giovan Paolo, all'interno di un provvedimento di legge comunitaria, che pare a sua volta un grande spreco

questo è il punto - potrebbero anche trovare un risanamento laddove venisse esplicitata la procedura, che invece nel testo dell'articolo 45 è solo evocata genericamente.

quindi non dando luogo ad una mera continuità tra i vecchi utilizzatori, proprietari e gestori delle frequenze analogiche (per tutti RAI e Mediaset), creando un'occasione per aprire una gara effettiva, e non con quello che nel gergo un po' di settore viene chiamato *beauty contest*, che gara - come sapete - non è; dà l'opportunità a nuovi soggetti di entrare, soggetti diversi da quelli che abbiamo conosciuto e che possono esercitare delle opportunità che il digitale, come nessuna altra tecnica, potrebbe loro garantire. È quindi fondamentale che il limite ai cosiddetti *multiplex* sia più rigoroso e che la possibilità per i nuovi entranti sia effettiva, che si calcolino anche i telefoni cellulari che entrano a pieno titolo dentro questo contesto, come sanno i più i più giovani che ormai stanno dentro l'universo cognitivo della rete più di noi adulti, e che vi sia un limite per la

un tema di questa portata, che riguarda il nuovo assetto del Paese per i prossimi 30-40 anni? Sarà questo il peso di un articolo siffatto? Non durerà pochi mesi, con il rischio peraltro di mantenere aperta un'infrazione comunitaria - non devo dirlo io a lei - e di impedire quel successo possibile di nuove opportunità comunicative e culturali? O lo stralcio, quindi, o un cambiamento profondo.

Lei sa quante persone, per esempio qui nel Lazio, ancora non sanno che il 16 giugno prossimo non vedranno più né RAI 2 né Rete 4, e che tra breve non vedranno più la vecchia televisione? Lo sanno

e che, dopo un veloce passaggio alla Camera, sarebbe stata pubblicata ed entrata in vigore in tempi brevissimi. Avevo allora espresso la soddisfazione per essere giunti all'approvazione del provvedimento, in quanto il ritardo che gravava sul testo, sfasato di più di un anno rispetto a quanto disposto al suo interno e rispetto anche a quanto recava il titolo «Legge comunitaria 2008», rendeva il provvedimento superato, e quindi era necessaria una veloce approvazione. Nella discussione in 14a Commissione ed in quella in Assemblea si era anche arrivati ad una sorta di compromesso, che aveva portato al voto favorevole dell'Italia dei Valori in quanto diversi dei nostri emendamenti ed ordini del giorno erano stati accolti. Mi riferisco, ad esempio, alla proposta sulla parità retributiva uomini-donne nel quale si chiedeva di impiegare le eventuali risorse liberate da una riforma del sistema pensionistico per gli interventi a sostegno dell'impiego femminile e dell'onere di cura familiare; familiare; erano stati accolti i nostri suggerimenti che chiedevano maggiori garanzie democratiche per gli stranieri condannati in Italia che con la decisione-quadro avrebbero scontato pene detentive nel loro Paese d'origine. Tutti questi motivi, nonché un generale convincimento che la legge comunitaria, con i suoi pregi e difetti, è un atto imprescindibile per assicurare che il nostro ordinamento sia conforme a quello degli altri Paesi europei hanno portato l'IdV a votare favorevolmente. Lo ripeto ancora: a determinare il nostro voto è stata anche la volontà di giungere al più presto ad un'approvazione definitiva del testo per non scadere davvero nel ridicolo di discutere ancora di un provvedimento relativo al 2008, mentre era già stato licenziato dal Consiglio dei ministri l'Atto relativo al 2009. Infine, voglio dirlo: il testo della legge comunitaria, così come si presentava nella sua versione originale, era stato originalmente redatto dal Governo precedente. Quindi, si trattava di un provvedimento frutto di un lavoro condiviso appieno. Diversa è invece la situazione che ci si presenta oggi dinanzi. Diversa quindi potrebbe essere la posizione dell'Italia dei Valori al momento del voto; anzi, sicuramente lo sarà. Innanzitutto, sono trascorsi tre mesi dall'approvazione in Senato, che rendono questo provvedimento ancora più anacronistico in quanto alla Camera il testo della legge comunitaria 2009 è stato già presentato in data 19 maggio, come Atto Camera n. La domanda da porsi, cari colleghi, è allora come sono stati impiegati questi tre mesi. Forse per accogliere i suggerimenti dell'opposizione? Forse per definire un provvedimento che si avvicina maggiormente a quanto disposto nelle direttive europee che si intende recepire o da quanto sancito dai princìpi generali comunitari, contenuti nei Trattati istitutivi di Comunità europea e UE? Non credo credo sia stato questo il motore che ha portato ad una modifica della legge comunitaria. Ritengo piuttosto che la vera ragione risieda nella volontà di utilizzare la normativa come un contenitore per inserire disposizioni che, purtroppo, risultano utili agli interessi di questo Governo. La discrezionalità con la quale il Governo, tramite i suoi emendamenti alla Camera, ha deciso quali norme europee recepire, come recepirle e quali invece escludere, dà conto di come nella maggioranza ci si interessi all'Europa soltanto se è una risorsa normativa valida per tutelare certi interessi o se è una scusante efficace per addossare colpe di inadempienze da parte del nostro Stato. L'operazione fatta è stata, in sintesi estrema, quella di uno *shopping* al supermercato delle leggi europee: questa legge sì, perché in favore delle categorie che voglio tutelare,

atteggiamento è il rifiuto di dare parere favorevole, impedendo quindi di integrarli nel testo, a dei validissimi emendamenti presentati dall'Italia dei Valori alla Camera. Penso, ad esempio, alla caccia. Nella legge comunitaria si deroga alla regolamentazione dell'attività venatoria, dando alle Regioni la possibilità di modificare il calendario contenente i divieti di caccia. di mantenere rigide regole che impedissero di effettuare la caccia nel periodo della riproduzione degli animali e di limitarsi per il calendario ad un semplice principio a cui le Regioni devono ispirarsi. Cari colleghi, già si violano le regole in Italia, figuriamoci i principi ispiratori. Tuttavia, l'emendamento non è stato accolto, forse perché gli interessi della *lobby* della caccia sono più forti e convincenti di quelli degli animalisti. esempio, cari colleghi, in cui il Governo ha scelto di tutelare gli interessi forti e non i soggetti deboli è in materia di qualità dell'aria. L'Italia dei Valori aveva chiesto di inserire lo standard della riduzione delle emissioni inquinanti del 20 per cento, così come richiesto dalla Commissione europea, ma purtroppo, ancora una volta, questa proposta Si sa che la forza dissuasiva dei produttori di auto e delle aziende industriali è incomparabile con quella dei cittadini con malattie respiratorie o di altro genere collegate all'inquinamento, ma lo Stato non dovrebbe tutelare proprio coloro che hanno forza contrattuale minore? Invece, nell'articolo 10 in questione, l'unica tutela che è stata prevista, con una bizzarra concessione fatta alla Lega, riguarda i cittadini della Pianura padana. Perché dovrebbero meritare più attenzione loro di coloro che vivono, per esempio, nei complessi industriali di Bari? Come glielo spiegano a quelli che si ammalano di tumore attorno alle fabbriche della Puglia? La risposta è la solita amara considerazione: valgono più gli interessi di potere e gli accordi fra partiti dell'alleanza di Governo che il bene pubblico. Ancora, per quanto riguarda la materia dei giochi di azzardo, come Italia dei Valori avevamo chiesto di inserire una norma che imponesse a tutti i circoli di poker privati che stanno nascendo e che stanno diffondendosi sul territorio

i circoli aprono come associazioni culturali e i giocatori d'azzardo che li frequentano, persone spesso affette da dipendenza psicologica da gioco, perdono miliardi di vecchie si rischiano tragedie di vite umane. Il Governo però preferisce tutelare chi con i circoli si arricchisce: camorra, mafia, 'ndrangheta. Ecco tutta una serie di provvedimenti che mostrano come davvero si scelga cosa inserire nella legge comunitaria sulla base di discrezionalità tutte proprie del Governo. Ma il caso più eclatante è quello della distribuzione delle frequenze radiotelevisive, e sul punto il senatore Pardi sicuramente farà una riflessione dopo di me. Mi riferisco al caso di Rete 4 ed Europa 7. Lo ripeto, con gli ordini del giorno che abbiamo presentato oggi in Commissione, come spiegheremo anche nel corso della loro illustrazione in Aula, si cerca di chiudere una procedura di infrazione già avviata dalla Commissione europea e di assicurare il pluralismo dell'informazione.

preannuncio che proprio su questo punto, per noi fondamentale, si deciderà come orientare il voto dell'Italia dei Valori. Vorrei sottolineare inoltre che, siccome ci è stato chiesto di non presentare una mole pesante di emendamenti, che avrebbe rimandato ancor più l'approvazione di una legge che oramai puzza di vecchio e che comunque avrebbe incontrato un'intransigente opposizione da parte della maggioranza, come Italia dei Valori abbiamo dimostrato la collaborativa responsabilità

in linea con le norme europee e con il nostro sistema di diritto. La legge comunitaria, dato il suo titolo e la sua natura, è una norma istituita per assicurare che la nostra Nazione rispetti il diritto e i principi della Comunità europea, fra cui figurano il pluralismo, la trasparenza e il diritto all'informazione. Cerchiamo di ricordarlo quando voteremo gli ordini del giorno dell'Italia dei Valori sulle frequenze televisive. Per inciso,

Dico questo pensando - con la preoccupazione, la rabbia e la tristezza che già ho manifestato pubblicamente, ieri e oggi, anche con il presidente Belisario- alla visita di domani di Gheddafi in questa che oggi approva la legge con cui si rispettano le norme europee, le quali domani però infrangerà insieme ai principi fondamentali dell'Unione europea, invitando un dittatore a parlare. Lascio a voi la risposta.

anch'io vorrei svolgere brevemente qualche considerazione preliminare, nel ricordare che questo nostro dibattito avviene dopo il voto per le elezioni europee. questa la sede e non abbiamo il tempo per l'esame di questo voto, ma credo che alcune brevissime considerazioni vadano fatte, soprattutto per le incognite

invece al dato che gli osservatori delle questioni europee ci hanno messo fortemente all'attenzione e che possiamo riassumere nell'aumento degli euroscettici come presenza all'interno del nuovo Parlamento.

di dirgli dove siederemo nel Parlamento europeo. Io credo che noi ci siederemo insieme alle forze della democrazia e del progresso

il partito di maggioranza relativa che sostiene questo Governo con il posto in cui siedono i suoi alleati principali, che si sono molto rafforzati in queste elezioni e che sulle questioni europee

quale sarà la politica rispetto all'Europa di questo Governo e della maggioranza che lo sostiene. Infatti, non solo noi, che possiamo essere come ci dite sempre - malevoli e pieni di pregiudizi, bensì tutti gli osservatori, analizzando la politica europea della Lega e quella del PdL (non parliamo di quella del Partito popolare europeo), notano delle differenze profonde.

Il processo con la Turchia, pur lento e graduale, vedrà la rappresentanza di questo Governo Governo seguirlo e portarlo avanti o subirà un blocco, come chiede, con coerenza e da sempre, la Lega? L'armonizzazione legislativa sul piano sociale e fiscale andrà avanti? punto non è questione di Lega o di PdL), rifaremo l'Alitalia nazionalista contro Air France per poi scandalizzarci di come va il rapporto FIAT‑Opel,

della politica estera del nostro Paese, di apertura di un ponte verso il mondo arabo, rafforzando la politica europea in questa direzione, oppure si crea, *extra* Europa, un canale privilegiato che avvantaggia solo qualcuno? Questa è un'altra questione che forse sarebbe interessante discutere, anche alla luce della circostanza di questi ultimi

care colleghe, cari colleghi, concentrerò il mio intervento (in meno dei dieci minuti che il Presidente mi ha concesso)

Come sappiamo, e come sottolinea la stessa direttiva al «considerando» n. 4, «i servizi costituiscono il motore della crescita economica»

di un mercato unico dei servizi in Europa, ma esso non deve andare a scapito della qualità dei servizi propri di ciascun Paese. È evidente che noi ci preoccupiamo della qualità dei servizi nel nostro Paese

trasparenza e di non discriminazione, tali da garantire il mantenimento o, se possibile, addirittura la promozione della qualità. Questi requisiti

è stata progressivamente elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del Trattato, e potrebbe continuare ad evolvere. La nozione, come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di giustizia, copre almeno i seguenti motivi: l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del Trattato, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertà di espressione dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessità di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria». Tutti questi sono considerati «motivi imperativi di interesse generale»

garantiscano la stessa qualità di prestazione legge comunitaria, all'articolo 41, comma 1, lettera *f)*, tra i princìpi e criteri direttivi

di carattere generale che possono essere utilizzati nella delega del Governo per l'imposizione di requisiti requisiti sono: ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente. Mi sembra veramente un po' poco. termini, la delega al Governo è più restrittiva di quanto la direttiva imponesse e a mio avviso ciò non è giustificato in ordine al principio base della direttiva stessa, sancito dall'articolo 1, che stabilisce la volontà di realizzare la libera circolazione dei servizi, mantenendo però costante la qualità dei servizi stessi. È importante che questo elemento venga

presentato alle pubbliche autorità. Tale firma ha dei riflessi importanti, in quanto ad essa corrisponde l'assunzione di responsabilità civili e penali

in essere delle disposizioni e dei requisiti affinché chi viene a prestare i servizi di ingegneria nel nostro Paese garantisca il mantenimento della qualità di tali servizi che nel nostro Paese è stata elevata. Ricordo che gli ingegneri nel nostro Paese debbono firmare gli elaborati di progettazione, direzione dei lavori e collaudo per una grandissima serie di opere. Mi sia consentita una loro breve enumerazione: edifici per abitazione civile e per uffici; strutture in cemento armato e in ferro per tali edifici; ponti stradali e ferroviari; gallerie; strade; vie ferrate; apparecchiature per il sollevamento di persone o cose; teleferiche e funivie; recipienti e tubazioni a pressione; impianti chimici; impianti petrolchimici; impianti manifatturieri; impianti elettrici; linee elettriche di trasmissione; dighe; condotte forzate; impianti termoelettrici; impianti nucleari (quando ci saranno); opere idrauliche; opere igienico-sanitarie (ad esempio i cimiteri); azioni di bonifica del territorio; macchine per il trasporto di persone e cose su strada; materiale ferroviario rotabile; aeromobili. Ecco, per tutte queste azioni l'ingegnere l'ingegnere si assume personalmente responsabilità civili e penali attraverso la firma di elaborati di progettazione, di direzione dei lavori e di collaudo. gli ingegneri che verranno a svolgere servizi di questo tipo in Italia abbiano la qualità che finora è stata garantita dagli ingegneri italiani anche attraverso norme deontologiche che

Signora Presidente, desidero ringraziare tutti coloro che hanno preso la parola in sede di discussione generale perché comunque, sia che abbiano espresso critiche al testo, sia che abbiano dato pareri favorevoli, hanno sicuramente fornito spunti di riflessione. Nello specifico, al

effettivamente stiamo vivendo un momento di incertezza riguardo al futuro dell'Europa;

esattamente se ci saranno cambiamenti nella linea di politica del mercato interno ed estero dell'Europa.

della tutela dei cittadini italiani nel recepimento della cosiddetta direttiva servizi è stato effettivamente compiuto. Andare al di là credo che ci avrebbe

abbiamo trasmesso l'idea forte che questo Parlamento ha comuni radici. Noi crediamo profondamente all'Europa, a questa opportunità importante. Penso che l'attività legislativa sia un treno fondamentale, un momento forte proprio per supportare ciò che diciamo con i fatti.

«La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea della Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, ad eccezione dell'articolo 33 sul quale il parere è di semplice contrarietà nel presupposto che il meccanismo di finanziamento dell'organismo ivi previsto sia posto a carico degli intermediari finanziari al fine di garantire l'assenza di oneri per la finanza pubblica. In merito agli emendamenti, esprime parere non ostativo».

Signora Presidente, l'emendamento 6.1 riguarda la modifica dell'*iter* delle nomine dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni, già citato dal senatore Di Giovan Paolo. Con tale emendamento si chiede di non citare i numeri totali della delegazione (la modifica introdotta dalla Camera), in quanto il Trattato di Lisbona, quando entrerà in vigore, assegnerà all'Italia più membri nel Comitato delle regioni di quanti ne abbia oggi. Quando il Consiglio europeo chiederà all'Italia di allinearsi al Trattato, il nostro Paese, se vigerà questo articolo non emendato, si troverà nell'impossibilità di adempiere velocemente

l'emendamento 6.1, tenendo fermo il principio generale della suddivisione della delegazione italiana tra autonomie regionali e locali, permette di gestire la materia in maniera più semplificata e veloce, proponendo di farlo attraverso un decreto del Presidente del Consiglio da approvare a seguito di intesa con la Conferenza unificata, com'è stato fino ad oggi ogni volta che si è dovuto procedere alla nomina dei membri ed alla loro surroga. Rappresentanti del Governo ed altri senatori che del Comitato delle regioni sono stati membri possono testimoniare che in quindici anni, da quando il Comitato delle regioni esiste, è sempre stato garantito il rapido svolgimento delle pratiche di nomina e, soprattutto, è sempre stata garantita la più ampia rappresentanza delle autonomie regionali e locali. signora Presidente, chiedo ai colleghi di sostenere questo emendamento, che va verso l'idea di una dialettica tra Governo e rappresentanti degli enti locali, di una semplificazione e soprattutto di una maggiore velocità delle procedure.

Grazie

È vero che si attende un riordino della normativa in materia, ma siccome questo articolo fa riferimento alla normativa europea, che è stata recepita, evidentemente gli alloggi nuovi dovrebbero soggiacere a tale normativa: del resto ciò già avviene in una serie di realtà. C'è però un altro problema, ovvero l'assoluta inapplicabilità di questo comma, perché si parla di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Signor Ministro, non esiste una definizione giuridica di questo tipo. Che significa «alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»? Si fa riferimento alla concessione edilizia, al verbale di ultimazione dei lavori, alla concessione dell'abitabilità degli alloggi?

A parte il merito, siamo davanti a un comma assolutamente inapplicabile dal punto di vista giuridico. Per questo abbiamo presentato l'emendamento, che sosterremo nel voto.

che era stata approvata all'unanimità alla Camera, che ripristina il divieto di somministrazione degli alcolici dopo le due di notte nelle discoteche. Esprimo la mia contrarietà perché penso che non si affronti un tema drammatico e anche tragico come quello della diffusione dell'alcool tra i giovani con norme di carattere proibizionista. In Senato c'è stato un accordo che ha coinvolto

alcune valutazioni che vanno nella direzione opposta a quella seguita dal collega dell'opposizione. Ringrazio invece il Governo che, accogliendo l'emendamento

che anzitutto riconferma la linea di questo Governo e della maggioranza che lo sostiene in ordine alla necessità di individuare criteri che non sono di carattere proibizionista, ma sono invece da iscriversi in un percorso legislativo, da inquadrarsi nella *ratio* che ispira tanto le norme che si stanno definendo sul pacchetto sicurezza quanto quelle relative al codice di educazione stradale. Tali norme fanno emergere il rapporto di stretta connessione tra l'utilizzo di alcool e gli incidenti; infatti, se si considera tanto la documentazione che abbiamo a livello nazionale quanto quella che ci proviene da fonte europea, si ha la triste conferma che una percentuale elevatissima di incidenti stradali è dovuta proprio al che il guidatore ha fatto uso eccessivo di alcool. Quindi, la norma, che peraltro era stata già licenziata in prima lettura da questa Camera, e poi inopinatamente modificata

che si intende destinare al problema, che troverà un suo completamento sotto il profilo della sensibilizzazione e dell'educazione dei giovani non soltanto al corretto utilizzo dell'alcool ma anche alla corretta conduzione di un automezzo. Ciò a riconferma dell'assoluta coerenza di questo provvedimento, che noi salutiamo con grande convinzione e con il massimo sostegno.

dell'argomento, per cui erano apparse un po' imprudenti e "incestuose" rispetto allo spirito dello strumento della legge comunitaria le incursioni avvenute alla Camera. Del resto, la mia proposta emendativa, proprio per la sua sobrietà, mi è sembrato abbia delineato un sentimento comune che lascia poi strade aperte per legiferare in un altro contesto. Di qui la mia gratitudine oltre che al Governo ai colleghi dell'opposizione.

l'emendamento 45.1 riguarda esattamente il tema di cui prima si è parlato, cioè il passaggio alla teca digitale. piacerebbe che questo emendamento venisse valutato per il suo valore di merito, al di là degli schieramenti politici. Forse è un'illusione, ma il mio suggerimento è di meditarci con questo testo forse si apre una strada diversa per il digitale in Italia.

Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non

come già lamentato in quest'Aula in occasione del voto in prima lettura lo scorso 17 marzo, la legge comunitaria che fa riferimento all'anno 2008 viene approvata dal Parlamento italiano con grande, colpevole ritardo. Abbiamo dunque più volte rilevato, nel corso dell'esame in Commissione, una preoccupante inclinazione da parte dell'Italia a subire procedimenti d'infrazione. Diverse sono, infatti, le procedure che rischiano tuttora di aggiungersi ad ulteriori sentenze di condanna, mediante le quali la Corte di giustizia impone anche sanzioni pecuniarie, che comportano pesanti oneri economici per le casse

I settori che sono oggetto del maggior numero di infrazioni sono quelli dell'ambiente, della fiscalità e degli appalti e riguardano soprattutto le carenze a livello regionale e locale. Le nostre proposte si sono concentrate in particolare sul tema della parificazione dell'età pensionabile tra uomo e donna. Abbiamo ritenuto opportuna l'introduzione del principio di flessibilità e volontarietà per la permanenza nel luogo di lavoro a favore di quelle donne che si sono impegnate nella cura dei figli o dei congiunti riconosciuti disabili gravi o dedite alla cura degli anziani. Con rammarico constatiamo che nulla di ciò viene previsto nel provvedimento che oggi il Senato approverà in via definitiva.

delle frequenze nel nostro Paese è puramente politica ed è evidente che l'elevato tasso di concentrazione del mercato televisivo italiano supera di gran lunga quello degli altri Paesi sviluppati. La legge comunitaria del 2008 non ha affrontato il problema centrale, ossia la garanzia di un vero pluralismo: in questo modo, si determinerà anche nel digitale una posizione di duopolio, già esistente nell'analogico. Ribadisco Ribadisco che il disegno di legge ritornato in Senato in terza lettura si ripromette di adempiere ad obblighi cui l'Italia avrebbe dovuto già da tempo La Camera ha approvato un certo numero di modifiche, tra le quali quelle della legge n. 11 del 2005 riguardante la nomina dei componenti italiani del Comitato delle regioni, il recepimento della normativa comunitaria in materia di inquinamento acustico, una lieve modifica riguardante la direttiva relativa alla qualità dell'aria in modo da garantire criteri omogenei sul territorio nazionale.

Positive sono infatti le norme a tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, appropriazione illegittima e imitazione, nonché quelle finalizzate finalizzate alla semplificazione amministrativa per gli adempimenti a carico dei produttori del settore del vino. Signora Presidente, cari colleghi, per i succitati motivi la priorità del provvedimento, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo.

che ho pronunciato tre mesi fa in quest'Aula, si chiudeva con una frase di Churchill, pronunciata nel 1946, dopo la Seconda guerra mondiale, nella quale si diceva che alla guerra intestina fra le Nazioni europee «esiste un rimedio che in pochi anni renderebbe tutta l'Europa libera e felice. Esso consiste nella ricostruzione della famiglia dei popoli europei, o di quanto più di essa possiamo ricostituire, e nel dotarla di una struttura che le permetta di vivere in pace, in sicurezza e in libertà». affermavo che l'Italia dei Valori, proprio per conseguire la pace, la sicurezza e la libertà, avrebbe votato favorevolmente alla legge comunitaria. Intendiamoci, questa nuova versione della legge comunitaria non è in contrasto con la pace, la sicurezza e la libertà, ma è in contrasto con alcuni princìpi fondamentali contenuti nei Trattati: trasparenza, pluralismo informativo, economia di mercato. Non mi stancherò di ripeterlo: le frequenze televisive e quelle digitali non sono un semplice strumento per l'esercizio di un'attività economica, ma sono anche mezzi che consentono, tramite la realizzazione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, di conseguire il diritto all'informazione. Ecco perché sostengo che se la legge comunitaria non va contro la pace e la sicurezza, va comunque contro princìpi parimenti importanti per ogni cittadino; che voi, giudicando le nostre proposte non nel merito ma valutandole solo nell'interesse autoreferenziale, avete purtroppo infranto. Per quanto riguarda il metodo con cui è stata gestita la discussione della legge comunitaria, vi sono dei vizi notevoli che non possono non essere denunciati: questa maggioranza ha bocciato i nostri ordini del giorno anche dopo che eravamo arrivati a un accordo, poi da voi infranto. Ci avete infatti chiesto di non presentare emendamenti, perché la legge aveva già un ritardo di un anno e mezzo sulla tabella di marcia

che non comportavano una nuova lettura alla Camera. E voi cosa avete fatto? Non solo avete bocciato gli ordini del giorno, ma avete approvato i vostri emendamenti;

La tesi è quella già ripetuta più volte: il Governo ha perso il senso del bene comune e persegue soltanto istintivi interessi personali.

accade per i trattati internazionali, sui quali, solitamente, il Parlamento vota a favore compatto. Ma la prassi che ci aveva visto agire sulla scena internazionale con decisioni *bipartisan* è cambiata.

poi redigendo leggi comunitarie di parte, come quella al nostro esame. Fa male, cari colleghi, fare questi discorsi a due giorni dalle elezioni europee. Dispiace di doversi dividere sulle disposizioni che dovrebbero ratificare norme europee, la cui iniziativa legislativa risiede nella Commissione europea e la cui approvazione è determinata dal voto del Parlamento europeo. Gli italiani sono andati a votare in massa per il Parlamento europeo, con una percentuale di partecipazione al voto di gran lunga superiore all'affluenza media europea. Gli italiani sono europeisti convinti. Sono più europeisti della maggioranza che li governa! Questo Governo decide di utilizzare la legge comunitaria come un menu *à la carte*, quando una direttiva comunitaria o una sentenza della Corte di giustizia vanno a vantaggio di un qualcosa che sta bene al Governo, allora vengono recepite,

non pensate forse che se l'affluenza alle urne, seppur imponente, è comunque diminuita di 6 punti percentuali rispetto alle elezioni questo sia dovuto alla semplice considerazione che ogni italiano avrà fatto, vale a dire: «Se all'Europa non danno importanza i partiti, i parlamentari, il Governo, perché dovremmo darla noi»? Dunque, questa legge comunitaria è un ennesimo tassello di quella mancata attenzione, che poi si traduce in euroscetticismo, in progressivo abbandono dell'esercizio del voto, in crescente distacco dalle istituzioni comunitarie.

mi perdonino i colleghi e soprattutto il ministro Ronchi - se ha un po' di accortezza e mi fa la cortesia di essere più attento

È anche per questo che ritengo non più ammissibile che anche la legge comunitaria, strumento legislativo per eccellenza ancora a cavallo tra l'ordinamento europeo e quello nazionale, diventi un coacervo di problemi e questioni che ne rallentano a dismisura l'approvazione. Un esempio evidente oggi è costituito dall'articolato sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche;

successivamente, alla Camera il Governo ha utilizzato un procedimento comunitario per mantenere inalterata la propria strategia in materia, guadagnando un anno sulla condanna certa della Corte di giustizia delle L'Italia è un caso unico nel panorama europeo e persiste nel voler rimanere un caso anomalo di deficit democratico. Tuttavia, nel parlare oggi di qualità e tempistica del trasferimento dell'ordinamento europeo in quello nazionale problema su cui abbiamo presentato un apposito ordine del giorno cui il Governo ha dato parere contrario - ci interessa affrontare la questione del voto europeo, che ha a che fare con il diritto comunitario ed è pertinente alla discussione odierna. Il risultato europeo è caratterizzato da un forte astensionismo, che non può essere considerato come un messaggio di indifferenza rivolto specificamente dalle opinioni pubbliche contro l'Europa. Il declino della partecipazione elettorale è un fenomeno che tocca ogni Paese europeo nella sua vita interna, tuttavia in questa tornata è opportuno sottolineare che all'insuccesso di partecipazione ha fortemente contribuito il carattere tutto nazionale delle campagne elettorali. Nel nostro Paese, inoltre, il carattere della competizione è stato condizionato anche da vicende create da una sola persona, che mantiene inalterata la confusione tra pratica politica privata e affari. Sul risultato nazionale, per quanto ci riguarda, non c'è nessun trionfalismo, ma è altrettanto evidente che il berlusconismo spinto ha fatto perdere consensi anche al Popolo della Libertà. Libertà. Dalla lettura europea dei risultati emerge un quadro in cui gli orientamenti dell'opinione pubblica appaiono uniformi, poiché ad essere penalizzate dal voto non risultano essere soltanto le forze socialiste e progressiste, ma in maniera meno vistosa anche le forze del centrodestra al Governo di 21 dei 27 Paesi membri dell'Unione europea. Siamo quindi in presenza di sintomi rivelatori di un'offerta politica povera, opaca, inadeguata al carattere europeo del voto. Torna quindi utile per questo ragionamento guardare alle forze che hanno registrato una certa espansione su scala europea, quelle che più di altre si sono situate in una dimensione politica sovranazionale, che sintetizzo in pro e contro l'unione politica e federale dell'Europa. In questi due campi, gli elettori hanno riconosciuto e ricompensato l'offerta politica più chiara e mobilitante. In questo stanno - a mio avviso - le ragioni di una riflessione seria che deve impegnare i grandi partiti europei, come recentemente evidenziato anche dallo stesso presidente del Partito popolare europeo, Wilfried Martens. Si sono infatti chiusi i riflettori della campagna elettorale ed è finito il tormentone sulla collocazione della delegazione del Partito Democratico, che non potrà che essere nel rinnovato campo dei progressisti e della sinistra europea. Il vero banco di prova è tutto nel campo del Partito popolare ed è rappresentato dalla intenzione dei conservatori britannici, cechi e polacchi di dare vita ad una destra euroscettica. Si tratta di una novità nello scenario politico europeo che implica una forte politicizzazione dell'Unione ed una ridefinizione dell'identità stessa del Partito popolare europeo per la naturale esigenza di far emergere le differenze come condizione di questa separazione. A questo punto il problema è dato dal sapere se il Popolo della Libertà, ma anche la Lega, sono pronti per una così urgente ridefinizione a livello europeo. di fronte ad una questione politica che ha a che fare con il futuro dell'Unione non si tratta solo di far valere i numeri, ma di verificare veramente la reale volontà la reale volontà di mettere in campo una forte convinzione europeista per sbarrare la strada a una destra nazionalista, e nelle sue frange estreme anche xenofoba. E, a proposito di numeri, è bene ricordare quanto tutto ciò abbia a che vedere con la coesione nazionale, come in più di un'occasione ha sottolineato il Capo dello Stato. Lungi, quindi, dal segnare una battuta d'arresto, le elezioni europee del 6 e 7 giugno, hanno impresso una forte accelerazione alla necessità di costruire uno spazio politico unificato europeo, perché i progetti più innovatori - la politica estera, di sicurezza e difesa comune, il voto a maggioranza nel Consiglio, le politiche economiche, sociali e sull'immigrazione, l'elezione diretta del presidente della Commissione - rischiano di restare incompiute finché non poggeranno su una democrazia costruita a misura europea. E chi dice democrazia, dice partiti, leader, capacità di costruire consenso. Solo offrendo risposte efficaci ai grandi problemi che ormai superano la capacità di azione degli Stati nazionali, l'Europa può riconquistare la fiducia e la passione dei cittadini. Tutto questo sta e stava nelle mani del Consiglio europeo, dominato dai Governi di centrodestra, che in questi anni hanno riportato a sé i veri poteri decisionali; mentre nel Parlamento europeo è il Partito popolare ad avere di nuovo la maggioranza relativa. E poiché il sistema di codecisione accresce le possibilità di veto parlamentare, il pericolo della paralisi legislativa è del tutto inesistente. Tutto ciò avrà un impatto fondamentale sul cammino verso sul cammino verso l'integrazione europea e accresce le responsabilità del Gruppo popolare europeo, in particolare delle delegazioni dei Paesi più grandi e, quindi, anche del Governo italiano. Richiamare questa realtà serve a sottolineare la difficoltà e la vera e propria povertà di collegamenti fra l'Italia e i vari livelli di governo europeo. Si tratta di un'anomalia formale che è opportuno rimuovere se si vuole contribuire a ridare autorevolezza e ruolo all'Italia nell'Unione. C'è urgente bisogno che il nostro Paese ritorni a essere protagonista del processo di costruzione dell'interesse comune, perché è soprattutto a partire da qui che si può poi ritrovare il giusto livello di mediazione per l'interesse nazionale. Vedete, colleghi, l'Italia oggi più di ogni altro grande Paese europeo ha tutto l'interesse ad adoperarsi per il rilancio dell'integrazione europea intesa come rafforzamento dei valori e delle politiche comuni. Occorre dunque collocare i problemi che interessano particolarmente i cittadini europei, come i temi della convivenza e dell'immigrazione, dove essi sono realmente: nel superamento dell'attuale debolezza politica dell'Unione di fronte alla crisi e alle spinte nazionaliste.

e la volontà di cooperare che abbiamo caparbiamente dimostrato nella nostra azione parlamentare fino all'ultima richiesta di stralcio della tematica radiotelevisiva,

e dell'Europa, non si possa prescindere da un reale pluralismo politico e culturale in grado di garantire trasparenza e concorrenza, valori oggi violati dall'Italia nel mercato radiotelevisivo europeo.

Onorevole Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi senatori, accogliamo questa legge comunitaria, in modo particolare per quanto attiene alle decisioni quadro adottate dall'Unione europea nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Mi riferisco alle norme in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, di scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri e di reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea. Ricordo ancora una volta che metà delle persone transitate per le nostre carceri nel 2007 era straniera (equivalente ad una spesa aggiuntiva di 7 miliardi di euro), che un reato su tre è commesso da clandestini, dei quali solo uno su nove, fra quelli identificati, viene realmente espulso. Grazie a questo provvedimento e alle successive norme e accordi internazionali volti a dar seguito ad esso, si potrà far scontare la condanna di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea nel Paese d'origine anche senza il consenso dell'interessato, attualmente obbligatorio per legge. Il Governo sta lavorando in questa direzione con l'adozione del decreto legislativo relativo all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali, senza dover attendere l'entrata in vigore della legge comunitaria 2009, che presumibilmente non avverrà prima dell'inizio del prossimo anno. Si tratta di un provvedimento che può costituire un ottimo deterrente per chi viene a delinquere nel nostro Paese, contando su un sistema carcerario decisamente meno duro rispetto a quello dei Paesi di provenienza. Quella di Bruxelles è una decisione quadro che dovrà essere recepita obbligatoriamente da tutti Paesi membri dell'Unione entro il 5 dicembre 2011, ma per quanto ci riguarda la situazione di emergenza criminalità che si è creata ha consigliato di accelerare i tempi; bisognerà poi solo attendere il recepimento della norma da parte degli altri Stati europei, per rispettare il principio della reciprocità. Nell'interesse comune ci aspettiamo, in particolare dalla Romania, fattiva collaborazione per rendere operativo l'accordo in tempi brevi. Il disegno di legge ritorna in Senato perché la Camera ha apportato un certo numero di modifiche, tra le quali le più importanti concernono la legge n. 11 del 2005 (disposizioni relative alla nomina dei componenti italiani del Comitato delle Regioni); disposizioni miranti ad evitare discriminazioni per i cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione; il recepimento della normativa comunitaria in materia di inquinamento acustico; lo stralcio integrale dell'articolo 16, che disciplinava la caccia; la soppressione dell'articolo 21 relativo alle bevande di fantasia; alcuni criteri di delega aggiuntivi per l'attuazione della cosiddetta direttiva servizi; l'attuazione, infine, della cosiddetta direttiva ricorsi in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Inoltre, ritengo importante sottolineare l'introduzione dell'articolo 43, che riguarda l'emergenza rifiuti in Campania, diretto ad abrogare un comma del decreto-legge n. 172 del 2008 che prevede un'autorizzazione comunitaria, non necessaria e non prevista, per l'individuazione dei siti di stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti, in attesa del funzionamento a regime del sistema dello smaltimento. Riteniamo che ciò consentirà di velocizzare l'*iter* burocratico relativo allo smaltimento dei rifiuti. In conclusione, dal lungo e tormentato *iter* del disegno di legge comunitaria 2008 emerge una necessità, quella di introdurre meccanismi di recepimento della legislazione comunitaria più snelli e razionali. L'euroburocrazia - e non l'Europa - è nel mirino del nostro movimento, perché si somma a quella - da noi ben conosciuta e che da sempre combattiamo - del sistema Italia, vecchia questione all'origine del nostro progetto di riforma federale dello Stato. Confermo comunque il voto favorevole al provvedimento in esame da parte del Gruppo Lega Nord Padania.

desidero anch'io sottolineare la felice circostanza che questa seconda lettura in Senato venga a coincidere con l'elezione del nuovo e rinnovato Parlamento europeo, che - non dimentichiamolo - è la nostra fonte primaria di ispirazione per quanto riguarda l'aspetto legislativo. Su questo ruolo, anche in questo dibattito, sono sorte perplessità e critiche; vi sono anche, a certi livelli, casi di rigetto, addirittura da parte di chi non intende riconoscere a livello comunitario una eccessiva invasività negli interventi legislativi e in tutti i settori di competenza dei Parlamenti nazionali. Mi si consenta un preambolo, ispirato proprio ai riflessi politici che le recenti elezioni europee avranno all'interno dell'Unione ed anche nei rapporti interistituzionali con i Paesi membri. Anche se prematura, la lettura dei dati è già possibile. Il dato politico - mi mi spiace per gli europessimisti - rassicura gli europositivi, cioè coloro che credono nel ruolo di coordinamento dell'Unione europea. Il voto infatti ha rafforzato notevolmente i gruppi tradizionalmente europeisti, come la grande famiglia dei popolari europei, dei socialisti, dei liberali, che sicuramente saranno coerenti nel loro impegno di rilanciare il processo di coesione e di integrazione nell'Unione europea. Non va però sottovalutata la presenza di nuove forze ispirate all'euroscetticismo ed anche a posizioni forse più oltranziste, che puntano al ritorno alle politiche nazionali. Stupisce, su questo terreno, anche qualche illustre personaggio, che non esita ad esprimersi. Il più famoso, soltanto una settimana fa a Parigi, è stato addirittura il presidente di turno uscente, il ceco Klaus, il quale ha manifestato tutto il suo europessimismo davanti all'assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale. Ebbene, Klaus probabilmente ha inteso in questo modo mascherare il totale fallimento del suo semestre di presidenza in Europa, aggravato anche da una crisi interna irreversibile. Queste forze critiche, di fronte a documenti tecnici di raccordo come questa legge comunitaria, non esitano a manifestare il loro dissenso. la massima considerazione e il massimo rispetto a questo tipo di visione dell'Europa, basata su una sorta di sospetto, di diffidenza, quasi di gelosia per presunti pericoli di esproprio di sovranità nazionale, fortunatamente assisteremo anche per i prossimi cinque anni ad un'evoluzione positiva dello spirito europeistico. su ventisette stanno facendo pressioni sull'Irlanda affinché accetti e recepisca il Trattato di Lisbona e dia via libera ad una serie di riforme indispensabili per favorire questa evoluzione europeistica. Il Trattato, che è solo una copia sbiadita della Carta costituzionale firmata a Roma nella primavera del 2004, accresce nello stesso tempo i poteri del Parlamento europeo nei confronti del Consiglio e dei Parlamenti nazionali nei confronti delle istituzioni europee. Il Parlamento europeo avrà nuovi spazi di codecisione; aumenterà anche il peso democratico dei cittadini europei. I Parlamenti nazionali si vedranno attribuire un ruolo nuovo e più incisivo nella fase di preparazione e di verifica dei percorsi legislativi su determinate materie. Importante è considerare queste riforme come un miglioramento delle condizioni del dialogo, non come una vittoria nel *derby* tra Parlamenti nazionali ed istituzioni europee.

perché presumibilmente e prevedibilmente la legislazione europea sarà più aderente alle esigenze e alle caratteristiche delle legislazioni nazionali. Come ha sottolineato la nostra eccellente relatrice Rossana Boldi, noi oggi voteremo solo sulle proposte di modifica pervenute dalla Camera dei deputati. Si tratta di ritocchi numerosi, ma non sostanziali, come è stato detto. In questo contesto, va sottolineata la volontà del Governo, manifestata in Commissione dal ministro Ronchi (che potrà ribadirla, se intende farlo, anche in questa sede), di favorire in futuro un *iter* più rapido più accelerato di questo passaggio, che consenta di consegnare la legge comunitaria al Parlamento nell'anno di esercizio e non, come accade oggi, a metà dell'anno successivo. E a questo proposito, sempre il ministro Ronchi ha annunciato di avere già incardinato la legge comunitaria per il 2009 presso la Camera dei deputati. Questo consentirà di recepirne le norme in tempi più rapidi rispetto alla tradizione italiana, che ci pone purtroppo agli ultimi posti nella classifica dei Paesi quanto al recepimento delle direttive. Il dibattito appena concluso ha già evidenziato molti aspetti che chiaramente non ripeterò. Il passaggio saliente, quello più dibattuto, riguarda l'articolo 23,

Si tratta della normativa relativa alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche, in relazione alla strategia comunitaria di riduzione, se possibile, dei danni derivanti dal consumo di alcolici, in merito alla sicurezza personale e in particolare a quella stradale. La Commissione del Senato ha infatti indicato nuovamente le ore 2 di notte come ora limite per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche. Particolarmente impegnata nella verifica del testo è stata la Commissione agricoltura: ricordiamo infatti che in Europa la politica agricola comune assorbe ancora oltre il 40 per cento del bilancio comunitario. Le modifiche proposte riguardano i settori del vino, dell'olio d'oliva, della grappa, delle bevande analcoliche a base di succhi di frutta e dell'allevamento avicolo. Il tenore delle osservazioni proposte parte dalla difesa della qualità, della salubrità e della tipicità delle produzioni come requisiti di mercato, ma anche come garanzia verso il consumatore, per passare poi alla trasparenza amministrativa, alla promozione e all'etichettatura. Per il vino, in particolare, l'articolo 15 - di cui ha parlato il collega senatore Pinzger - chiede di irrobustire il regime comunitario che garantisce le denominazioni di origine e di indicazione geografica per migliorare la competitività dei prodotti e rafforzare la riconoscibilità dei vini italiani sui mercati esteri. Ciò a garanzia dei produttori, oltre che come difesa contro le contraffazioni. Anche nel settore delle bevande alcoliche, della grappa in particolare, l'articolo 17 introduce severi disciplinari per assicurare standard di qualità garantiti ed evitare contraffazioni. Per l'olio d'oliva l'articolo 17, comma 2, impone l'indicazione in etichetta dell'origine geografica, come garanzia ancora una volta di di genuinità e di conformità alle normative europee, ma anche alle tradizioni italiane di qualità. Per le bevande analcoliche a base di agrumi, c'è l'imperativo di garantire che il contenuto di agrumi non sia non sia inferiore al 12 per cento. Una particolare attenzione è stata posta alla salute animale: l'articolo 37, al comma 9, stabilisce norme per l'allevamento delle galline ovaiole, ma anche per garantire la salubrità del prodotto.

di trattamento dei cittadini italiani, rispetto agli altri cittadini europei, in rapporto al recepimento delle norme europee. Lo spirito degli adeguamenti di cui ho parlato è quello di difendere la particolarità delle esigenze nazionali, ma sempre nel contesto comunitario, quindi senza farsi mettere i piedi in testa - siamo d'accordo - ma senza rimettere ogni volta in discussione la nostra appartenenza all'Unione europea, che ci ha garantito, tra l'altro, 60 anni di tranquillità, di pace e di progresso.

"per effetto della crisi l'immagine popolare dell'Europa è diventata un po' dappertutto meno asettica, meno dogmatica, più empirica e questa evoluzione è positiva.

una crisi biblica come questa in condizioni tutto sommato di competitività. Insomma, l'Europa si può mettere in discussione, si può criticare tutti i giorni, ma non le si può voltare le spalle, quindi annuncio il voto favorevole

oggi il signor Beppe Grillo, in audizione presso la 1a Commissione affari costituzionali, tra le altre affermazioni, ha dichiarato quanto segue. «Questa Commissione, questo Parlamento non hanno nulla a che fare con la democrazia. Sei persone hanno deciso i nomi di chi doveva diventare deputato e senatore, hanno scelto 993 amici, avvocati e qualche zoccola e li hanno eletti». Il signor Beppe Grillo non si può permettere di delegittimare gratuitamente la rappresentanza femminile al Senato. Non può ergersi a giudice parziale contro tutte a prescindere, colpevolizzando a tappeto i membri del Senato, come se lui fosse l'unico santino puro e casto. A nome di tutte le colleghe senatrici, informo la Presidenza che tutte ci sentiamo profondamente lese nella persona e nel ruolo che ricopriamo, donne di maggioranza e di opposizione; che ricopriamo con serietà e dedizione, altro che zoccole! Annunciamo la nostra querela per diffamazione avverso il signor Beppe Grillo.

Presidente, il nostro Gruppo contesta questa sua decisione per la semplice ragione che non si è mai visto che in fase di voto finale si dia la parola - seppure per ragioni assolutamente condivisibili

non me ne voglia, ma lei ha palesemente violato una decisione assunta dalla Presidenza del Senato che noi avevamo accettato, pur se modificava una prassi che era molto più garantista nei confronti di tutti i componenti dell'Assemblea; che questa sua decisione non costituisca un precedente.

Dichiaro aperta la votazione.

Sospendo la seduta per venti minuti.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo

il Senato non è in numero legale

Colleghi, posso chiedere un momento di silenzio? La Presidenza deve rendere delle comunicazioni all'Aula prima del voto finale.

Onorevoli colleghi, la Presidenza del Senato ha appreso, con stupore e rammarico, delle dichiarazioni rese nella giornata odierna dal presentatore di un disegno di legge d'iniziativa popolare, Beppe Grillo, in occasione di un'audizione presso la 1ª Commissione permanente. Nel condividere le considerazioni critiche e ferme della vice presidente della stessa Commissione, senatrice Maria Fortuna Incostante, la Presidenza, con riserva di valutare ulteriori seguiti della questione, respinge con forza le espressioni volgari di insulto rivolte ai rappresentanti eletti dal popolo.

Non ci si può rivolgere al Parlamento e, nello stesso tempo, offenderne i componenti. L'offesa volgare e qualunquistica delle istituzioni è uno strumento già usato, con esiti drammatici, nel corso della storia del nostro Paese. Sì, quindi, alle critiche, ma forte deve risuonare il nostro no alla volgarità ed alla delegittimazione preconcetta delle istituzioni rappresentative. È nostro dovere saper cogliere quanto, a volte con asprezza, chiede a noi la pubblica opinione. Mai però dobbiamo assecondare istinti e pulsioni che nulla hanno a che fare con la necessaria riforma e la tutela delle istituzioni democratiche della nostra Repubblica.

Non ho né l'intenzione, né il compito di difendere quanto è stato detto da Beppe Grillo. Osservo di sfuggita che la riunione della Commissione solo a tratti ha avuto i connotati istituzionali tipici dell'esposizione di un disegno di legge, di una motivazione e di domande da parte dei parlamentari presenti. Probabilmente,

si ponga il problema di intervenire giudicando lo stile del comportamento adottato da un audito. Ho trovato corretto il comportamento della presidente Incostante, che ha fatto capire all'audito che doveva esprimersi in maniera diversa, ma mi sembra abbastanza curioso che l'intera Aula assuma un compito di giudizio su espressioni stilisticamente scomposte. che però mi colpisce ancora di più è che la stessa severità analitica e di giudizio sulle espressioni non è stata usata in altre occasioni di rilievo straordinariamente superiore. Non posso dimenticare che il Presidente del Consiglio, non un presentatore televisivo, ha più volte detto, ribadito e ripetuto in varie sedi, pubblicamente e con linguaggio altrettanto stilisticamente scomposto, che il Parlamento è fatto da persone che stanno lì a votare in massa senza sapere cosa fanno e che nel Parlamento forse sarebbe meglio votassero solo i Capigruppo.

e allora tanto più deve assumere tale atteggiamento critico quando le parole scomposte sono...

che si può liberamente giocare con le parole, allora si prendono anche le conseguenze dell'uso del lessico. Anche il Presidente del Consiglio è un parlamentare e quindi noi, a tutto diritto, potremmo considerarlo il cappone di Palazzo Chigi.

Signora Presidente, ho chiesto la parola sullo stesso argomento che ha affrontato il senatore Pardi perché fui oggetto di una vivacissima e - mi permetto di dire - anche scomposta reazione

della Camera. Mi permetto di dire che, al di là di ogni questione lessicale, dobbiamo stare molto attenti a censurare sempre e ogni volta, da chiunque provengano, affermazioni che riguardano la legittimazione del Parlamento e la sua funzione, perché altrimenti ci indeboliamo noi per primi e ci esponiamo a osservazioni come quelle che oggi il dottor Grillo ha fatto in 1a Commissione nel corso della sua audizione.

l'essenza stessa della democrazia), non possiamo farlo una volta sì e una volta no a seconda di chi parla. Questa non è materia di polemica politica, questa è materia che sta oltre. Sono tanto più forte oggi nel rigettare le affermazioni fatte dal dottor Grillo in 1a Commissione, peraltro anche nei confronti delle componenti di Camera e Senato, in quanto sono capace di difendere i componenti di quest'Aula e il lavoro del Parlamento sempre, altrimenti è ovvio che non disponiamo più di nessuna arma ed è questo l'errore grave in cui è caduta la maggioranza nell'occasione che ho ricordato poc'anzi. Mi lasci anche dell'inappropriatezza con la quale la Presidenza del Senato ha, in quell'occasione, affrontato la questione e ha reagito Oggi mi pare che si sia adottata la reazione giusta; non è possibile però avere due registri, perché i valori in gioco sono esattamente gli stessi

Signora Presidente, onorevoli colleghi, crediamo che la tutela dell'immagine e dell'onorabilità di chi svolge la funzione di senatore ed è impegnato nel

avremmo gradito che la stigmatizzazione fosse condivisa da tutti i Gruppi politici, senza alcuna esitazione, perché non è ammissibile in questo settore applicare il principio, come ho sentito dire poco fa, della compensazione delle colpe. Se c'è stato un errore, non è possibile accettare che questa colpa vada a compensare una colpa che è quella commessa oggi dal cosiddetto dottor Grillo in Commissione affari costituzionali con un'accusa specifica e volgare,

pur essendo stato condannato con sentenza definitiva per omicidio colposo, per aver ucciso due persone adulte e un bambino di otto anni. *(Applausi dal Gruppo LNP).* Non ci è mai passato per l'anticamera del cervello di usare espressioni di questo tipo. Eppure questa persona oggi ha usato quella espressione. Nessuna compensazione di colpe, Per noi questo è un fatto gravissimo e tale lo abbiamo definito e qualificato. Signora Presidente, colleghi senatori, la storia del parlamentarismo è tutta segnata da un confine che separa la critica legittima dalla denigrazione delle istituzioni parlamentari. Non tutto può essere qualificato come antiparlamentarismo e la critica al funzionamento del Parlamento, alla razionalità è parte integrante del parlamentarismo stesso e della sua storia. Lo è, per quel che ci riguarda, dalla storia della Costituente. Per chi conosce la vicenda del parlamentarismo lo è da secoli, ed espressioni anche più colorite di quelle che sono state utilizzate dal Presidente del Consiglio le ritroviamo in ogni pagina degli atti dell'Assemblea costituente,

che si debba confondere; non credo lo si debba fare perché si commette un errore. Voler catalogare tutto indistintamente sotto la voce

limpida, su quelle dichiarazioni c'è stata una legittima critica da parte delle opposizioni alla quale si è replicato dando il senso di che cosa quelle espressioni significavano. Evidentemente il dissenso rimane, ma rimane nell'ambito di quella fisiologia di cui è fatto il confronto tra maggioranza e opposizione. Non mi sembra francamente che si possa mettere sullo stesso piano il turpiloquio che è stato oggi udito in 1a Commissione. E non lo si può fare a maggior ragione perché quella di oggi, l'audizione dell'"onorevole" Grillo, era una libera concessione che questo Parlamento aveva fatto nei confronti di una iniziativa popolare, chiamando in qualche modo al suo interno coloro i quali questo Parlamento lo criticavano con quella iniziativa, quindi dimostrando la superiorità delle istituzioni rappresentative e la loro capacità inclusiva. Non vorrei francamente che qualsiasi cosa venga riportata nello stesso schema e che qualsiasi avvenimento diventi comunque un modo per criticare direttamente o indirettamente il Presidente del Consiglio. Questa è ossessione, non libera critica, e secondo me è un atteggiamento sbagliato. Dobbiamo semplicemente constatare che in quella occasione c'è stato un libero dibattito, che ci ha visto divergere. Oggi, ciò che dovrebbe risultare, di fronte a quelle dichiarazioni, è invece che

ha nutrito i nostri dibattiti e non la abbandoniamo. Non ci stanchiamo di proporre in ogni occasione, e non strumentalmente, critiche al funzionamento di questo Parlamento, allo scopo di migliorarlo, e non permettiamo che queste critiche siano confuse con le offese che abbiamo ascoltato oggi.

una scelta un po' illogica e irrazionale. A fronte dell'irrazionalità di questa modalità di inviare il segnale audio nelle cabine degli interpreti, mi chiedo anche chi ha fornito quei pannelli e chi ci sarà nelle cabine per le traduzioni. Come diceva qualcun altro, a pensar male si farà pure peccato, ma spesso ci si azzecca. Visto che che spesso noi adottiamo dei sistemi di sicurezza importandoli a volte dalla Cina ‑ e non vorrei che domani o anche oggi li abbiamo importati dalla Libia ‑ mi chiedo e chiedo alla Presidenza che cosa sono. La seconda domanda è la seguente: il cerimoniale di domani cosa prevede?

Signora Presidente, intervengo anch'io su alcune questioni che sono in qualche modo collegate al tema Libia. Non affronterò la questione della giornata di domani; altri sono intervenuti su questo aspetto. Vorrei semplicemente sottolineare un tema e mi dispiace che non ci sia più nessun rappresentante del Governo; lo segnalo comunque alla Presidenza e chiedo che rimanga agli atti di questa seduta. Da tre legislature attende una soluzione il problema delle imprese creditrici della Libia. imprese che sono state espulse a suo tempo da quel Paese e che hanno vantato crediti che non sono ancora stati onorati. Il Trattato di amicizia che è stato ratificato in quest'Aula

che possono concorrere alla soluzione del problema. C'è un *gap* fra i 450 milioni riconosciuti dai libici ‑ come ci ha detto il ministro degli affari esteri Frattini ‑ e i 650 milioni vantati dalle aziende italiane. Devo dire che qualcuna ha già risolto

Credo che sia molto importante tutto quello che accadrà (insieme ai problemi che sono stati sollevati), ma questa è una questione concreta che dovrebbe essere avvertita come un dovere istituzionale

e insopportabile che dalla prossima settimana - o da quella successiva - noi in Commissione non fossimo in condizione di chiudere una questione che rappresenta veramente un'ingiustizia assoluta, a maggior ragione in presenza di un

Signora Presidente, faccio mio quest'ultimo intervento del senatore Barbolini. Per i cultori della materia - la materia sarebbe quella di onorare un dittatore - ricordo che domani sera, alle ore 21, su Sky verrà trasmesso il film «Il leone del deserto», un film che nel 1982 era proibito in questo Paese perché recava danno all'immagine e alla reputazione delle nostre Forze armate. Oggi che abbiamo finalmente al Governo la maggioranza del Popolo della Libertà, che vorrebbe mettere l'Esercito dappertutto, credo che sia significativo che, tra le varie onorificenze che vengono attribuite e riservate a Gheddafi, ci sia anche questa. La seconda notizia è che per acclamazione - perché non si fanno mancare nulla nemmeno alle Nazioni Unite - oggi è stato eletto presidente dell'Assemblea generale libico per gli affari africani Ali Triki. Questo signore, nei mesi scorsi, aveva lanciato una campagna nei confronti dei Paesi dell'Unione africana, che qui verrà rappresentata (anche se speriamo di no, perché magari in questo preciso istante si sta discutendo in Conferenza dei Capigruppo di adottare una decisione di tipo diverso), di tipo diverso), volta a indurli a ritirarsi dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, perché il loro fratello Al Bashir era stato incriminato per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Lo ripeto: perché noi, o magari le «truppe cammellate» che verranno importate in quest'Aula domani mattina qualora decidessimo di non essere presenti, dobbiamo concedere il diritto di tribuna a tutto ciò che ho elencato (e non si tratta che degli ultimi sviluppi di una situazione che va avanti da 40 anni)? Con la senatrice Poretti siamo in sciopero della fame o, per meglio dire, in digiuno di dialogo con la Presidenza del Senato, da stamani. Il digiuno non è che uno degli strumenti della non violenza politica: c'è la non collaborazione, c'è la disobbedienza civile e c'è comunque la pratica delle proprie convinzioni. Questo è un ulteriore spunto di riflessione per la decisione che in questi minuti si apprestano a prendere in Conferenza dei Capigruppo, in relazione alla riunione di domani mattina alle ore

un dittatore in Aula, e dal momento che si concede di far piantare una tenda faraonica al dittatore Gheddafi a Villa Pamphili, giardino pubblico e bene culturale, non capisco perché il Gruppo dell'Italia dei Valori il Gruppo dell'Italia dei Valori dovrebbe "alzare le tende" dall'Aula del Senato, nella quale rappresentiamo ogni giorno l'interesse dei cittadini italiani che ci hanno democraticamente eletti. Crediamo di averne più diritto noi del dittatore libico: per questo annuncio sin da ora che intendiamo, come Gruppo, rimanere in Aula ad oltranza,

i diritti umani, per i clandestini che sono stati utilizzati come merce umana. Aspettiamo e, fino ad allora, non ci muoveremo dall'Aula.